Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo riunitasi oggi pomeriggio ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 16 luglio. In relazione alla richiesta della 5a Commissione permanente di poter disporre di più tempo per concludere l'esame del decreto-legge sulla manovra economica, le sedute di domani non avranno luogo. Con l'intesa che non potranno esservi ulteriori proroghe per la Commissione, la discussione del provvedimento da parte dell'Assemblea avrà inizio inderogabilmente giovedì mattina alle ore 9,30 e proseguirà nel pomeriggio e venerdì mattina, nonché la prossima settimana nelle sedute di martedì 13 e mercoledì 14, al fine di pervenire alla votazione finale entro la seduta pomeridiana di mercoledì 14 luglio. Il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea è stabilito per le ore 18 di domani. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi secondo il prospetto riportato in allegato al calendario, al fine di assicurare un ampio ed approfondito dibattito. Si ricorda la convocazione del Parlamento in seduta comune giovedì 8 luglio alle ore 14,30 per l'elezione di otto componenti del CSM. La chiama inizierà dagli onorevoli senatori. Per quanto riguarda il prosieguo dei lavori della prossima settimana, a conclusione del decreto-legge sulla manovra economica, a partire dalla seduta antimeridiana di giovedì 15 luglio sarà esaminato il decreto-legge in materia ambientale e di autotrasporto, già approvato dalla Camera dei deputati. Per la discussione del provvedimento sono previste sedute con votazioni anche nel pomeriggio di giovedì 15 e, se necessario, nella mattina di venerdì 16 luglio. Nei prossimi giorni la Presidenza ricorderà le figure di tre ex senatori recentemente scomparsi: Pietro Milio, giovedì 8 luglio alle ore 9,30; Rina Gagliardi, martedì 13 luglio alle ore 11; Egidio Sterpa, giovedì 15 luglio alle ore 9,30. Dopo gli interventi della Presidenza, potranno intervenire i rappresentanti dei Gruppi per 5 minuti ciascuno. La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre stabilito che nella seconda metà del mese di luglio saranno esaminati documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Infine, su richiesta di alcuni Gruppi, il Governo ha assicurato che renderà comunicazioni alla Commissione competente sulla situazione dei profughi eritrei in Libia.

di arrivare ad una migliore rappresentatività delle organizzazioni sindacali e ad una normativa sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro che rafforzi il *referendum* e l'efficacia dei contratti collettivi di lavoro.

lavoro e l'efficacia dei contratti collettivi. Molte volte ci siamo chiesti cosa può fare, in tempo utile, la politica per aiutare le vertenze più difficili; ebbene, il Senato potrebbe

torno in quest'Aula sulla vicenda, delicata, e in qualche modo anche simbolica, della fabbrica FIAT di Pomigliano Si è svolto, come tutti sanno, il *referendum* sull'accordo stipulato tra la FIAT e la maggior parte dei sindacati. Pomigliano, la sua vicenda, il suo dramma, nei giorni scorsi, ha avuto anche una grandissima attenzione mediatica; ora che che l'attenzione mediatica si è spenta, vorremmo sollevare qualche preoccupazione e chiedere al Governo una parte attiva almeno in questa fase. La preoccupazione è che, finita la grande attenzione per la vicenda, anche un po' simbolica e originale che si è svolta in quella fabbrica,

in cui siano rappresentate le parti, affinché, per prima cosa, la FIAT confermi l'investimento senza i se, senza i se, i ma ed i forse di questi ultimi giorni. La finalità del tavolo dovrebbe essere poi anche quella di un allargamento dell'area del consenso da parte del sindacato e dei lavoratori, anche al di là di quel 63 di definire, signor Presidente, in quali condizioni vivranno i lavoratori di quell'azienda in questo anno e mezzo di transizione, prima cioè che l'investimento diventi concreto. Ci chiediamo

Senatrice Armato, la Presidenza prende atto della sua richiesta. Ovviamente, se lo ritiene, può anche presentare un'interrogazione sull'argomento. **Per la

riguardante la misteriosa morte di Niki Aprile Gatti, che fu arrestato e venne trasferito a Firenze, nel carcere di Sollicciano. Si è trattato di uno stranissimo suicidio, e la mamma chiede ragione e giustizia.

parcheggiata l'auto a lato della strada, si gettava dal cavalcavia di via Cilea nel quartiere del Vomero a Napoli, morendo sul colpo. Tutti e due strani suicidi, per i quali i familiari chiedono giustizia.

31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, in corso